A conclusione dell'informativa, l'Aula riprenderà la propria attività alle ore 16,30, come già previsto dal calendario definito la settimana scorsa. Per l'esame del decreto-legge in materia di immigrazione i tempi sono stati ripartiti tra i Gruppi secondo lo schema riportato in allegato al calendario.

Verranno esaminati il bilancio interno e il rendiconto del Senato, l'eventuale seguito di argomenti non conclusi, il disegno di legge di modifica dello Statuto del Fondo monetario internazionale, nonché le ratifiche di accordi internazionali definite dalla Commissione affari esteri. È stata inoltre richiesta la disponibilità del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti a rendere un'informativa sul recente incendio avvenuto presso la stazione ferroviaria di Roma Tiburtina. Dopo la sospensione per la pausa estiva, le Commissioni potranno convocarsi a partire da lunedì 5 settembre. L'Assemblea L'Assemblea tornerà a riunirsi martedì 13 settembre, alle ore 16,30, per l'esame dei disegni di legge recanti rendiconto e assestamento del bilancio dello Stato. Nel corso di tale settimana, sarà convocata la Conferenza dei Capigruppo per stabilire gli altri argomenti da inserire nel calendario dei lavori.

mio Gruppo e gli altri Gruppi di opposizione non hanno ritenuto di votare questo calendario, per una ragione che è tutta e squisitamente politica, e che vorrei esporre brevemente Da qualche settimana il Parlamento è impegnato nell'esame di provvedimenti molto importanti, direi assolutamente importanti per definire l'affidabilità del nostro Paese e delle sue istituzioni, nonché la tenuta complessiva delle istituzioni, anche rappresentative.

sui mercati finanziari un'aggressione all'Italia tra le più virulente che la nostra storia ricordi. Oggi, il Parlamento è impegnato nella discussione del provvedimento sulle missioni internazionali, su cui si è già svolta

e unanime approvazione del disegno di legge, fatto salvo ovviamente quello che accade sempre tutte le volte che si affrontano provvedimenti di questo contenuto, che sono provvedimenti che sollecitano la coscienza individuale dei colleghi. Nella Conferenza dei Capigruppo della settimana scorsa, tra i provvedimenti pronti per l'esame dell'Aula, era stato elencato anche quello intitolato «Modifiche agli articoli 438, 442 e 516 e introduzione dell'articolo 442‑*bis* del codice di procedura penale. Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo». Il testo, già licenziato dalla Camera, originariamente recava all'articolo 1 la previsione della inapplicabilità del rito abbreviato ai reati puniti con la pena dell'ergastolo. Ma questo contenuto non esiste più,

la non utilizzabilità ai fini della prova del fatto accertato in altro procedimento con sentenza passata in giudicato. Credo che rientri tra i molti provvedimenti che hanno suscitato, nel Parlamento e nel Paese, un conflitto aspro e direi definitivo, in quanto attiene alla radice delle volontà orientate alle modifiche del codice penale e del codice di procedura penale; ma, tra i tanti provvedimenti, questo è uno di quelli che si segnala per la sua straordinaria gravità. Non può sfuggire a nessuno di noi

Mi chiedo se siamo nelle condizioni di poter affrontare uno scontro di questo genere. Non parlo soltanto a nome del mio Gruppo: parlo davvero a nome di questa e dell'altra Assemblea rappresentativa, avendo sentito anche i colleghi dell'altro ramo del Parlamento (comunque rappresentiamo i due Gruppi più consistenti di Camera e Senato).

Chiedo che questo provvedimento venga eliminato dal calendario e che venga rinviato in Commissione, perché si possa tornare ad un più meditato esame

anche se non in quest'ordine naturalmente, con l'esame del decreto‑legge in materia di rimpatri.

La prima ragione riguarda la circostanza che ci troviamo ad esaminare un provvedimento, quello che riguarda il cosiddetto processo lungo, che secondo noi, ai sensi del primo comma dell'articolo 97 del Regolamento, è improponibile. Infatti il testo esaminato dalla Commissione riguarda solo ed esclusivamente un oggetto specifico e predeterminato: l'inapplicabilità del rito abbreviato ai delitti punibili con la pena dell'ergastolo. Il testo licenziato dalla Commissione ha cancellato i cinque articoli che disciplinavano il rito abbreviato con riferimento a questi questi delitti ed ha introdotto due disposizioni che nulla hanno a che vedere, né dal punto di vista sostanziale, né da quello formale, con l'unica modifica al codice di procedura penale che riguarda questo aspetto del rito abbreviato. È stato infatti introdotto l'obbligo dell'ammissione delle liste testimoniali su istanza di parte in maniera assolutamente automatica ed è stata prevista peraltro l'introduzione di una norma transitoria, disposizioni ad una serie predeterminata e sospetta di procedimenti in corso. È stato inoltre scardinato uno dei principi fondamentali del nostro ordinamento giuridico, che riguarda la cosa giudicata. di disposizioni che con il testo approvato dalla Camera ed esaminato dalla Commissione non hanno nulla a che vedere e che quindi secondo noi, a norma dell'articolo 97 del Regolamento, non possono trovare ingresso e discussione in quest'Aula. Questa è la prima considerazione. La seconda considerazione è che questa mattina la Commissione affari costituzionali ha dato il parere sul decreto rimpatri, il cui esame, a mio avviso, dovrebbe essere anticipato.

sulla questione legata alle espulsioni. Noi stiamo modificando sostanzialmente la disciplina relativa al trattenimento degli irregolari nei centri di identificazione, di identificazione, introducendo un regime di custodia cautelare preventiva senza che si sia in presenza di un reato vero e proprio, e lo stiamo facendo senza avere alcun dato rispetto alle modalità e alle espulsioni, a quanto sta avvenendo nei centri di identificazione e rispetto anche

ammazza-processi e il decreto sui rimpatri entro giovedì mattina, perché questi sono i tempi di esame e di dibattito. In un giorno e mezzo,

Ora, signor Presidente, sostanziale del codice di procedura penale, in alcune parti particolarmente importanti, il che significa cambiare il processo penale e la dinamica del processo penale. Dovremmo modificare il sistema di trattenimento degli irregolari nei centri di identificazione, equiparandoli a coloro che si fanno sei mesi di custodia cautelare in carcere per delitti che sono di gravità superiore dal punto di vista del disvalore sociale e ordinamentale, rispetto alla permanenza irregolare nel nostro Paese. E tutti questi argomenti dovremmo approvarli in un giorno e mezzo.

il suo richiamo è pertinente, ma non cambia, mi consenta, il contenuto del mio intervento, perché noi abbiamo sì sedute di Aula fino a giovedì prossimo, ma la seduta della prossima settimana che noi, eventualmente, dovremmo dedicare dovremmo dedicare ad argomenti non conclusi consiste in mezza giornata. Quindi, da un giorno e mezzo

sia più giusto trattare l'ordine di priorità secondo altre esigenze; comunque, proprio per le ragioni che lei illustrava, se noi disponiamo di qualche giorno in più, non vedo la ragione per la quale dovremmo concludere entro giovedì questi due argomenti, a maggior ragione nel momento in cui possiamo esaminare il decreto-legge che riguarda i rimpatri, essendo stato questo esaminato dalla Commissione ed essendo a scadenza, e nonostante il rifiuto della maggioranza e del Governo di farci

come correttamente lei ha ricordato, alla seduta precedente, bensì alle modalità ed ai tempi di esame dei provvedimenti che erano stati già inseriti all'ordine del giorno, visti la loro complessità ed i loro profili di improponibilità a norma del Regolamento. Presidente, colleghi, cercherò di usare toni garbati anche considerando

dall'altro c'è stata un'autentica furbata nel mettere in calendario un provvedimento con un oggetto

dalla presidente Finocchiaro, né le argomentazioni del presidente D'Alia. Voglio ricordare a me stesso e, se consente, a lei e all'Assemblea che il 12 e 13 giugno il Paese, con milioni di voti, ha detto un no secco a nuove leggi personali per il Presidente del Consiglio. Invece, il Parlamento continua ad essere sequestrato per approvare norme che nulla hanno a che vedere con la riforma complessiva della giustizia.

i rapporti tra maggioranza e opposizione, che abbiamo cercato di mantenere su un profilo di gradimento istituzionale - come abbiamo dimostrato la settimana scorsa - andranno inevitabilmente a degradare, perché questo provvedimento è veramente l'ennesima vergogna agli occhi del Paese. Presidente, un provvedimento delimitato e circoscritto, che senz'altro avrebbe potuto essere condiviso dal Senato

di «Inapplicabilità del giudizio abbreviato per il delitti puniti con l'ergastolo» si è nel frattempo trasformato, come è capitato tante volte nel corso di questa legislatura, ed è diventato un organismo, non so se geneticamente modificato, ma considerevolmente modificato, e assume oggi una diversa denominazione, che leggo: «Modifiche agli articoli 438, 442 e 516 introduzione dell'articolo 442-*bis* del codice di procedura penale. Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo». Ovvero, è diventato l'ennesimo provvedimento *ad hoc* per porre mano a precisi procedimenti giudiziari. È evidente che l'opposizione non può dare il suo assenso a questa prospettiva. Mi associo quindi alle considerazioni dei colleghi dell'opposizione e, da ultimo, a quelle del senatore D'Alia, ha ricordato come una materia complessa come quella di cui al decreto rimpatri, che ha termini cogenti e può essere portato all'attenzione dell'Aula per la sua conversione, vada affrontata e approvata con le eventuali modifiche prima di questa controversa normativa. Ci opponiamo al calendario interverremo al momento giusto affinché venga ristabilita questa priorità logica, politica legislativa. Non possiamo, su queste basi, concordare con il calendario delle ultime due settimane. Aggiungo qualcosa che probabilmente susciterà qualche

passare con procedure troppo rapide il processo lungo: non si addice ad un processo lungo un procedimento parlamentare troppo breve, perché il provvedimento troppi aspetti relativi allo svolgimento delle attività giurisdizionali del nostro Paese. Come è capitato altre volte, per risolvere alcuni problemi si rischia di complicarne infiniti altri. È un film che abbiamo visto troppe volte e non possiamo aderirvi.

inserito all'ordine del giorno all'unanimità nella scorsa riunione, è stato approvato in Commissione tre mesi fa

pazientemente atteso. Quindi, nessun *iter* breve per questa norma, anzi un *iter* molto lento e approfondito in Commissione e una lista di attesa lunghissima, posto che sono passati diversi mesi dalla sua definitiva approvazione in Commissione e che la sua indicazione per l'Aula ha gli stessi contenuti, che adesso alcuni

di posizioni. Vorrei capire qual è l'oggetto della discussione, posto che quel calendario è stato approvato all'unanimità e, quanto a quello della settimana prossima, si vuole non discutere il bilancio?

la Presidenza aveva riconosciuto un fatto sostanziale, e cioè che le lagnanze, le censure dell'opposizione erano di carattere politico più che procedurale perché, appunto, il calendario era stato approvato, la Presidenza aveva già dichiarato che non si sarebbe sottratta dal consentire doverosamente ad ogni Capogruppo di opposizione di manifestare in quest'Aula la propria posizione, cosa che naturalmente è stata garantita, e che sono pronto a ripetere, perché il tema è squisitamente politico. Cionondimeno, siccome la Presidenza cercherà, si sforzerà di gestire questi passaggi delicati che ci porteranno alla conclusione dei lavori la prossima settimana con estrema cautela ed attenzione, anche per cercare di non disperdere il clima al quale faceva riferimento il presidente Belisario nel suo intervento, che ci ha portato ad approvare la manovra di bilancio nel giro di tre giorni, in un clima di grande assunzione di responsabilità, premesso che la vicenda tocca temi squisitamente politici, a me sta il compito e la funzione, complicata ed estremamente delicata, di fare in modo di non disperdere quella coesione politica e parlamentare che abbiamo registrato nei giorni trascorsi in occasione dell'approvazione della manovra.

di assumere delle iniziative coinvolgendo i Capigruppo per la prosecuzione dei lavori che toccheranno i futuri temi.

non di conflittualità, ma di rispetto delle regole. Vi posso garantire che le regole le rispetterò, ma cercherò anche di mediare per arrivare ad un clima di confronto e non di scontro.

apre una nuova finestra"), *segretario*. «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sul testo, con le seguenti condizioni, formulate ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione: all'articolo 5, sia inserito, in fine, il seguente comma: "7. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica"; - all'articolo 10, comma 1, la parola "escluso" sia sostituita dalle seguenti: «esclusi l'articolo 3, con la seguente osservazione: - per quanto riguarda i commi 9, 10 e 11 dell'articolo 3 - relativi alle modalità di gestione delle risorse non impegnate nell'anno finanziario di competenza - si raccomanda, in futuro, una più scrupolosa aderenza al principio contabilistico della destinazione In relazione agli emendamenti, la Commissione esprime parere di nulla osta sulle proposte 1.2, 2.12, 2.13, 4.3 e 6.3, aventi tutti una copertura sul Fondo per gli interventi strutturali di politica economica (FISPE) con l'intesa che, qualora tutte le proposte fossero approvate, dovrebbe essere verificata la capienza del Fondo ai fini della congruità delle coperture. Esprime poi parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 2.1, 3.1, 3.103, 4.105, 4.0.1, 4.0.3, 4.0.4, 4.0.5, 4.0.6, 4.0.7, 5.0.1, 5.0.2, 6.101, 8.1,

vale peraltro l'osservazione relativa a tutti gli emendamenti che trovano copertura sul FISPE. Infine, esprime parere di semplice contrarietà sull'emendamento 1.4. Il parere è di nulla osta su tutti i restanti emendamenti ad eccezione che sugli emendamenti 6.2 (testo 3), 4.1 e 4.0.2, sui quali il parere è sospeso».

sugli emendamenti 4.1 (testo 2) e 4.0.2 (testo 3), mentre, in relazione all'emendamento 6.2 (testo 3) esprime parere di nulla osta a condizione che, alla lettera c), primo periodo, siano soppresse le parole: "entro il 15 dicembre 2011" e le parole: "fino a tale data". Esprime altresì parere di semplice contrarietà sull'ultimo periodo dei medesimo emendamento. Si osserva inoltre che, poiché gli emendamenti 1.2, 2.10, 2.1.2, 2.13, 4.3 e 6.3 trovano tutti copertura sul Fondo per gli interventi strutturali di politica economica (FISPE), si intende che il parere su tali emendamenti sia contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, qualora gli emendamenti approvati

di mantenere la nostra presenza sui teatri più importanti (non soltanto quelli ai quali si riferisce la recente decisione della comunità internazionale di mandare delle truppe per garantire la pace e la stabilità internazionale, sia che si tratti dell'egida delle Nazioni Unite, sia che si tratti dell'Unione europea

Ci sono poi questioni che credo non possano non essere prese in considerazione, e che purtroppo si ripresentano ogni qualvolta ci troviamo di fronte al rinnovo del finanziamento delle missioni italiane all'estero. Mi riferisco al fatto che questo decreto è diventato

in esame distrae l'attenzione, includendo nella possibilità di finanziamento anche interventi

dei fattori e che, se anche non fa cambiare il risultato dal punto di vista economico, se non altro per pudore sposta l'accento sulla parte militare piuttosto che su quella

Le questioni più grandi, che avrebbero dovuto far dichiarare inammissibili alcuni emendamenti, per estraneità di materia, riguardano in del valore di 16.700.000 euro che noi diamo ad un Paese in cui, a mia memoria, non è stato sparato un colpo, in termini di conflitto internazionale, dalla Seconda guerra mondiale ad oggi, cioè Panama. Andiamo poi a finanziare con 60.000 euro un Centro di studi italo-tedesco, "Villa Vigoni", dove tutto si studia tranne che le missioni internazionali, i problemi relativi ai Paesi in via di sviluppo o le istituzioni internazionali che dovrebbero sancire la presenza dei vari contingenti nel mondo: lo si deduce anche da una rapida visione del sito Internet, dalla quale si deduce anche che al contempo questo istituto è sito in luogo favoloso, bellissimo. Quindi, si capisce magari anche perché si è deciso di includere qui dentro, tra l'altro appianando un debito che l'Italia si portava avanti, questi 60.000 euro. Si continuano a dare 300.000 euro a semestre all'Iniziativa adriatico-ionica, i cui prodotti un giorno saremmo curiosi di vedere. Se ne erano dati nello scorso semestre ad un altro fantomatico istituto, il cui sito Internet era aggiornato ad un anno e mezzo fa. Oggi si continua a dare danaro ad una iniziativa che dovrebbe parlare di grandi strategie per l'area adriatico-ionica, ma che almeno al Parlamento non si degna neanche di far sapere quel che fa.

Noi vorremmo che queste persone fossero accasermate nelle strutture di pertinenza del Ministero della difesa: questo sicuramente sarebbe uno dei

chiamiamola così - di passare tutte le ore di dibattito sia in Commissione sia anche negli incontri avuti con i Ministri degli affari esteri e della difesa,

9 affida al Ministero della difesa la riduzione del numero dei nostri militari presenti in tutto il mondo: prima 1.000 - ci è stato spiegato che erano quelli a bordo della "Garibaldi" - e poi altri 1.070, che non ci è stato spiegato da dove verranno presi (mi pare che questo non sia mai emerso). Se uno dovesse fare la somma di tutte le piccole missioni, lasciando fuori Afghanistan, Libano, Libia, Iraq e Balcani,

affida al Ministro della difesa la possibilità di chiudere venti presenze italiane nel mondo. Ciò che noi avremmo voluto con questi emendamenti, ma che avremmo ancor più voluto se si fossero rispettati gli impegni all'inizio dell'anno, quando, attraverso un ordine del giorno del senatore Di Giovan Paolo e altri senatori, si era arrivati a decidere che, prima di introdurre questo tipo di provvedimenti, avremmo dovuto svolgere un ampio e approfondito dibattito relativamente alla qualità, oltre che alla quantità, delle nostre presenze nel mondo. scenari - e mi avvio alla conclusione - in cui continuare per inerzia - parlo soprattutto della nostra piccola presenza - sicuramente non dà niente dal punto di vista qualitativo al mandato di tali missioni, ma ve ne sono altri, penso in particolare particolare all'Afghanistan e alla Libia, dove, se non si torna a parlare di politica e a fare delle proposte politiche, la mera presenza o azione militare non riuscirà, come purtroppo non sta riuscendo in quei due fronti, a portare a casa né la sicurezza, né la pace internazionale. L'Afghanistan ancora una volta sulle prime pagine dei nostri giornali perché un altro italiano è morto l'altro giorno, e ce n'è un altro purtroppo in fin di vita. Siamo diventati ormai specialisti esclusivamente nel cordoglio, ma non si recupera mai un'idea politica che sia una. La zona dove sono caduti i nostri militari è di massimo transito di sostanze che sono poi utilizzate per la produzione della droga, al ritorno ci si passa con le armi. Ecco, di fronte ad una crisi umanitaria come quella della Somalia, dove oltre al cibo ci sarà bisogno di analgesici, occorrerebbe un attimo fare mente locale, e magari prendere in considerazione la proposta fatta più volte - che il sottosegretario Crosetto ci ha addirittura detto essere stata fatta in parte proprio anche da questo Governo - di trasformare quell'oppio in analgesici. Per quanto riguarda la Libia ne parleremo più avanti, quando si arriverà all'ordine del giorno relativo all'articolo 2. Quindi, signor Presidente, la sollevo anche dall'incomodo di chiedermi tutte le volte se voglio illustrare gli emendamenti, perché con questo mio intervento li ho illustrati,

si rende necessario per aumentare l'importo da erogarsi per le iniziative e gli interventi di cooperazione a favore dell'Afghanistan, indicati sia al comma 1 ma anche ai successivi, sottraendo risorse al significativo incremento di spesa a favore della missione militare nello stesso Paese.

insegnare e per educare alla sanità, non per tenere un'arma in mano e morire all'interno di mezzi che tutto sono meno che che sicuri per la vita dei nostri militari (di questi, infatti, 41 purtroppo hanno perso la vita). Questo è un emendamento per riflettere sulle situazioni e sulla condizione che i nostri militari vivono in un ambiente che non è

i nostri militari allo sbando, perché è di sbando che bisogna parlare: persone che non sono preparate, che non hanno un adeguato non hanno un adeguato addestramento, di questo abbiamo già discusso nelle altre occasioni. Abbiamo ricordato non solo i morti, ma anche il nostro no fermo e convinto ad un finanziamento che non appartiene al nostro Paese. Su tutti questi argomenti gli emendamenti volgono alla seguente riflessione:

ne scaturisce che la metà della somma, chi è di 16 milioni e mezzo, per l'esattezza 8 milioni, viene coperta nella prima fase con i fondi del Ministero degli esteri, e quindi con tagli, peraltro flessibili. C'è l'impegno del Governo - in tal modo rispondiamo anche ad una richiesta complessiva emersa in sede di Commissione con proposte di emendamenti - a che la parte che in questo momento viene anticipata

di come si possa fare. In realtà, nella restituzione sarà compreso l'aumento di 8 milioni, che complessivamente era stato concordato in Commissione. Pertanto, politicamente c'è la conferma di quanto era stato deciso in Commissione. C'è la conferma peraltro dell'esigenza di un accordo precedente di mantenere i saldi di detta operazione. Quindi, con questo movimento di copertura andiamo politicamente a rispondere a quanto avevamo convenuto in Commissione. Nel dire che il Governo si esprime favorevole desidero spiegare che la stessa risposta vale anche per gli emendamenti proposti all'articolo 2.

parecchie imprese italiane, sia che abbiano lavorato in Libia sia che abbiano lavorato come subappaltatrici in Italia, hanno subito il rischio Paese e il rischio commerciale. Già ad Abu Dhabi si era stabilito in un gruppo di contatto la possibilità di scongelare i fondi

Nell'ordine del giorno è inserita anche una parte più strettamente finanziaria, perché chiediamo anche che le scadenze fiscali per le suddette imprese possano essere prorogate al momento dell'incasso dei crediti.

Signor Presidente, colleghi, colgo l'occasione di illustrare l'emendamento 2.14, che pone una questione di impegno da parte del nostro Paese nel Corno d'Africa e che mi auguro

precisare che anche chi di noi non ha partecipato al voto sulle missioni nelle precedenti occasioni, non ha mai voluto non partecipare al lavoro di costruzione di un modo diverso di presentare le missioni internazionali.

È il modo migliore, o potrebbe essere uno dei modi, per chiarire con certezza una politica estera e di sicurezza e difesa del nostro Paese che appartenga a tutti, al di là delle posizioni. Soltanto dopo si farebbero le scelte su quali missioni prendere in considerazione, ad esempio su questioni che emergono come questa del Corno d'Africa. La seconda questione riguarda - lo dico con molta chiarezza - la relazione con la cooperazione. Credo che debba esserci una differenziazione tra il lavoro di cooperazione e il lavoro delle missioni militari.

chi è non violento - lo dico anche al Ministro della difesa, perché su questo abbiamo fatto delle riflessioni - sa benissimo che non bisogna essere imbelli. La non violenza è diversa dal pacifismo *tout Allora, eliminiamo la retorica patriottarda e anche quella antipatriottarda. Essere non violenti vuol dire porsi la questione di come reagire a situazioni concrete. Nella ex Iugoslavia morirono nostri militari, nostri cooperanti e obiettori di coscienza,

Abbiamo bisogno che sia così, forse anche fornendo truppe all'Unione europea e alle Nazioni Unite. Questo pensa chi è non violento: non di mettere da parte o di porsi il problema di eliminare i rischi, ma di fare scelte rispetto a questo. un'altra questione, che è collegata a questo argomento, e per cui ritiro l'emendamento 7.100 (testo 2), che riguarda la scriminante sulla questione dell'eccesso colposo di legittima difesa. Vorrei essere molto chiaro su questo

quanto significa che dovremo confrontarci sulla politica estera e di sicurezza e difesa, come la chiamiamo in Unione europea; significa fare scelte anche per noi che aspiriamo ad essere un Governo alternativo al vostro, che alcune missioni dovremo farle e dovremo dire quando, come e dove, anche noi che siamo non violenti. È una sfida che facciamo prima di tutto a noi stessi, ma quell'articolo 9 significa che l'ordine del giorno di cui ero primo firmatario, sottoscritto anche da altri colleghi, va tradotto in pratica: dovete venire qui, e sulle oltre 30 missioni dovete dire come andiamo avanti e come

2011 e sopprimendo le parole «nel territorio da esso effettivamente controllato», perché ricordo che il riconoscimento del CNT da parte del Governo italiano è come unico legittimo rappresentante del popolo libico (quindi è meglio non fare precisazioni sui territori controllati).

dello IAI ne abbiamo parlato mille volte in Commissione. Che ora si venga in Aula facendo finta di non sapere cosa è lo IAI, francamente... Comunque, personalmente sono disposto ad invitarla a cena e a spiegarle cos'è lo IAI, e come lo IAI abbia ottenuto dal Consiglio europeo del 23 giugno il riconoscimento della macroregione europea adriatico‑ionica, perché riguarda l'area dei Balcani, dove mi pare che un problema di stabilità sia comunque alla nostra attenzione.

facendo presente che, sulla situazione specifica del Corno d'Africa e sulla Conferenza regionale, come ho avuto occasione di dire in Commissione, siamo in una fase estremamente delicata. La rappresentante speciale dell'ONU pensa di organizzare una Conferenza a Mogadiscio entro la metà di settembre. In questo momento, al di là di accogliere un ordine del giorno, e di intervenire

credo che leggerla in Aula sarebbe un esercizio non produttivo. L'altra scuola di pensiero, la mia personale, è che quando un ordine del giorno viene così profondamente modificato, è giusto dire che non viene accolto.

posto che accetto l'invito a cena del sottosegretario Mantica, e poi pubblicheremo il conto sui nostri siti Internet, per parlare dello IAI, si sa che cos'è ma non si sa cosa faccia

stata avanzata anche dalle Commissioni riunite con l'emendamento 3.3. Chiediamo di sopprimere i due commi che prevedono l'eliminazione delle figure dei volontari e dei cooperanti previsti dalla legge 26 febbraio 1987, n. 49, legge che regola la disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo. Non comprendiamo per quale motivo all'interno di un decreto-legge di rifinanziamento delle missioni internazionali sia stata introdotta tale riforma del sistema della cooperazione (il decreto, come sappiamo, va a rifinanziare l'operatività del secondo semestre dell'anno 2011). Questa previsione normativa, che con l'emendamento a mia prima firma si intende sopprimere, disarticola la cooperazione, compromettendo la continuità dei progetti già approvati e finanziati dal Ministero degli affari esteri, intervento che giunge - è utile ricordarlo - a seguito di una serie interminabile di tagli al settore in questione, mentre centinaia di migliaia di euro continuano ad essere assegnate a non meglio specificate iniziative ioniche e adriatiche dalla dubbia utilità, e milioni di euro vengono stanziati al fine di garantire la mancata cessione di unità navali alla società che se l'era aggiudicata, il tutto per adempiere ad un impegno preso con Panama. Anche sotto il profilo della qualità della legislazione, il Governo in questo caso dà riprova ancora una volta di capacità davvero illimitate. di approvare l'emendamento in questione, il quale prevede anche una ampissima copertura finanziaria data dalla soppressione del comma 1 del successivo articolo, riguardante la missione militare in Afghanistan, in modo che con tanti finanziamenti i progetti davvero di cooperazione possano trovare la concreta attuazione. Mi affido quindi all'Assemblea, certa del voto favorevole.

in gioco la missione in Afghanistan. Quanto all'emendamento 3.3, approvato dalle Commissioni riunite su nostra richiesta, abbiamo chiesto che venisse tolta dal decreto una norma che ridefiniva i rapporti amministrativi tra il Ministero e le organizzazioni non governative di volontariato internazionale. Abbiamo chiesto al Governo di ritirare la norma perché non ci sembrava questa la sede giusta

il comma che si intende sopprimere riguarda la missione in Afghanistan, iniziata nell'agosto 2003 in ambito ISAF, dove l'Italia, anche per coprire errori di strategia altrui, partecipa con un numero considerevole di uomini e di mezzi. Nel secondo semestre dell'anno sarà operativo nel teatro afgano un contingente stimabile in 4.200 unità. Il precedente decreto di proroga aveva previsto una totale di 3.790 unità, con un'ulteriore aggiunta di 180 unità a partire dal 1° novembre 2010. Secondo quanto previsto dal decreto-legge in esame, al comma 1 dell'articolo 4 è autorizzata, dal 1° luglio al 31 dicembre 2011, la spesa di quasi 400 milioni di euro per la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni ISAF Afghanistan, 20 milioni in più del semestre precedente. Occorre ricordare che il Consiglio dell'Unione europea ha istituito, con l'azione comune 2007/369/PESC del 30 maggio una missione PESD denominata *European Police Afghanistan* (EUPOL Afghanistan) alla quale l'Italia partecipa con il compito di favorire lo sviluppo di una struttura di sicurezza afgana sostenibile ed efficace, in conformità agli standard Sono trascorsi nove anni dall'inizio della nostra presenza in quella regione e i risultati sono sotto gli occhi di tutti: i talebani sono sempre più forti, il traffico di droga è aumentato, i signori della guerra si sono arricchiti, dando vita a sultanati indipendenti, la corruzione regna sovrana, le elezioni sono state inficiate da brogli di ogni genere, come è stato certificato da organismi internazionali, le donne e i bambini sono sempre in pericolo costante. Appare acclarato ormai che la missione di pace, sia essa di *peace-keeping* o di *peace-enforcing*, alla quale era stato destinato il nostro contingente ha prodotto un fallimento, e ciò va ammesso in ragione del fatto che tale missione ha in maniera evidente cambiato la propria natura nel corso del tempo trasformandosi in presenza militare, in violazione dell'articolo 11 della Costituzione; va segnalato, in tal senso che, per le sole missioni ISAF ed EUPOL, il nostro Governo ha stanziato, dal 2002 a oggi, oltre 3 miliardi di euro, dei quali circa il 90 per cento destinati per armamenti e equipaggiamenti e solo il restante per interventi di carattere civile, quindi di ricostruzione e aiuto alla popolazione. Gli attentati, sempre più frequenti, ai danni non solo dei militari italiani impegnati in Afghanistan mostrano chiaramente che il livello della potenza devastante degli esplosivi utilizzati dai ribelli talebani si è elevato; parallelamente, le dotazioni in uso dei nostri militari risultano al momento non più adeguate. Va, infine, ricordato che il 2010 è stato l'anno più sanguinoso da quando i talebani sono stati cacciati, con il contributo delle forze degli Stati Uniti e delle forze afgane, tant'è che è stato pagato un tributo in termini di militari pari a circa 750 uomini e donne, tra i quali i nostri. Per questi motivi, riteniamo che i nostri militari debbano tornare a casa, perché non possono stare lì a combattere una guerra non loro, sotto il falso vessillo delle missioni di pace.

Considerato che comprendo bene la ragione per cui non dobbiamo scrivere che si tratta di una disposizione in favore dell'aeroporto di Trapani, anche se sappiamo tutti che è così,

al finanziamento dei 10 milioni di euro. L'espressione «sentite le Province» significa sostanzialmente che il Ministero adotta il decreto senza che la Provincia interessata svolga

pensare di coinvolgere ancora meglio il sistema delle autonomie locali. (*Applausi vorrei segnalare il malfunzionamento del mio apparato di voto nella prima votazione

«si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie relative alle spese rimodulabili

che sono conseguentemente accantonate e rese indisponibili fino a concorrenza dell'onere. A questo scopo si applica quanto previsto dall'articolo 10, comma 14, del decreto legge n. 98 del 2011, in materia di flessibilità nella gestione del bilancio». Con questa copertura, gli

che è stato poi riformulato dal relatore e che ampiamente soddisfa le attese dei territori in cui vi sono state limitazioni ai voli civili a causa della risoluzione ONU 1973, ritiro tutti gli altri emendamenti a mia firma. Ringrazio il relatore ed il

5.1 fa riferimento alla necessità di inserire nel testo del comma 1 dell'articolo 111 del codice dell'ordinamento militare

il subemendamento 5.100/1

imbarcare sulle navi dei *team* militari o servirsi di agenzie di sicurezza private, quindi delle guardie giurate.

obblighiamo gli armatori e le agenzie di sicurezza italiane che hanno regolare licenza ad assumere soltanto degli italiani: questo contrasterebbe con la normativa europea, che invece consente la libera circolazione anche dei lavoratori, e sarebbe foriero di una infinità di ricorsi.

l'emendamento 6.5, come riportato dalla scheda di lettura del Servizio studi, elimina un riferimento al decreto-legge n. 228 del 2010 che non corrisponde ad alcuna disposizione del decreto stesso.

Presidente, in realtà l'emendamento 6.3, che sempre con il collega Totaro avevo presentato, era volto a rimpinguare le dotazioni riferite alle necessità di reclutamento delle Forze armate, in particolare dei volontari di truppa nelle loro varie accezioni, che erano state fortemente ridotte a seguito dei noti

alla stessa questione ed è stato elaborato sulla scorta delle proposte iniziali di chi parla e del senatore Totaro. Seppur con

come residui negli anni successivi, e in particolare nell'esercizio 2012, i fondi destinati all'intervento a favore delle vittime di malattie contratte nelle nelle missioni e in siti in cui i militari siano stati esposti a particolari rischi. Per semplicità lo chiamiamo emendamento uranio, ed è stato condiviso in sede di Commissione anche

al Ministero di completare alcune procedure per il riconoscimento di una sorta di cause di servizio che, a seguito delle lungaggini, non si è potuto completare nel termine dell'assegnazione dei fondi a ciò destinati. Penso si tratti di un intento condiviso dalla stragrande maggioranza dei parlamentari,

per la contestazione di reati molto gravi alla criminalità organizzata e ai terroristi. Ora, l'emendamento in questione non ha assolutamente nulla a che fare con il testo del provvedimento che stiamo esaminando, il quale già dal titolo indica indica questioni completamente diverse. Come ben sappiamo, il decreto‑legge in esame parla di interventi di cooperazione allo sviluppo, di sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, di missioni internazionali,

particolare e sensibile della nostra storia, in piena epoca di terrorismo e di criminalità organizzata. Esso tende ad introdurre soprattutto due norme che noi riteniamo estremamente gravi,

luogo non c'entra nulla; in secondo luogo, è pericoloso; in terzo luogo, costituisce un segnale politico negativo che la politica darebbe al Paese. Quindi, in prima battuta, signor Presidente, le chiedo che venga dichiarata l'inammissibilità di questo emendamento aggiuntivo.

riteniamo che sia perfettamente ammissibile all'interno del provvedimento in esame, anche perché riguarda i criteri per distinguere le armi di carattere militare, riservate alle Forze armate e ai corpi militari armati dello Stato, da quelle comuni da sparo. intendiamo neanche prendere in considerazione qualsiasi tipo di accostamento demagogico e assolutamente assurdo fra questo tipo di emendamento e quanto è successo in Norvegia. Non c'è proprio nessuna forma di attinenza, nessun elemento che possa

La legge n. 110 del 1975 è stata fatta proprio per fare chiarezza sulle armi detenibili dai cittadini, introducendo i criteri per distinguere le armi di carattere militare da quelle comuni da sparo. Tale funzione è venuta meno a seguito dell'approvazione di una legge altrettanto importante, la legge 9 luglio 1990, n. 185, che ha definito con chiarezza tutte le armi da considerare come facenti parte del materiale d'armamento e quindi escluse dalla legittima detenibilità da parte dei cittadini. È venuta meno quindi l'esigenza di distinguere le armi militari da quelle comuni, ed è venuto meno il senso del catalogo nazionale delle armi comuni da sparo, previsto dall'articolo 7, di cui oggi proponiamo l'abrogazione, della legge n. 110 del 1975. Il catalogo, come oggi viene applicato, costituisce anche una chiara violazione del diritto comunitario e sulla questione, senatore Perduca, è stata sollevata una procedura d'infrazione comunitaria, perché la normativa sul catalogo viola l'articolo 12

oggi che sottoponiamo una questione per la quale già esiste una procedura d'infrazione comunitaria che porterà a breve ad una condanna del nostro Paese, veniamo accusati di qualsiasi tipo di nefandezze. Ecco perché riteniamo che l'emendamento sia perfettamente ammissibile e chiediamo che l'Assemblea l'approvi.

alle caratteristiche di sicurezza e alla possibilità di vendita delle armi che il Parlamento ha votato nel recepimento della direttiva. Le norme inserite, che valgono per tutti i Paesi dell'Unione,

normativa vigente, riportato anche nel diritto comunitario, e semplicemente mantiene la classificazione degli istituti nazionali di prova, che certificano una per una le armi, come avviene in tutta l'Unione europea, rispetto alla possibilità che queste vengano messe in commercio. Altro non toccato dall'articolo è la rigorosa normativa italiana sulla legittimazione alla detenzione, all'acquisto e all'uso che appartiene al diritto domestico di ogni singolo Stato. Perché questo articolo e perché le Commissioni riunite - mi risulta tra l'altro con voto unanime - ne hanno consentito l'inserimento? Perché questo orpello, cioè il catalogo nazionale, che non ha più senso, è composto da una ventina di consulenti e funzionari, che oggi interverrebbero a valle rispetto alla classificazione che in tutta Europa - e oggi finalmente anche in Italia - viene fatta dagli istituti di banco di prova, che realizzano le verifiche sulle singole armi. Il risparmio di questi 20 consulenti e di questo desueto meccanismo, che costa diverse centinaia di migliaia di euro all'anno, è una delle risorse finanziarie dalle quali attinge il provvedimento in esame per consentire di disporre di ulteriori fondi per la manutenzione e l'approvvigionamento dei militari presenti nelle missioni di pace. È quindi una razionalizzazione coerente con il diritto comunitario, che mantiene un livello di sicurezza e di rigorosità, come avviene nel nostro ordinamento, rispetto all'acquisto legittimo delle armi da fuoco e alla loro commercializzazione e mette a disposizione risorse, oggi pagate dalle aziende, che verranno destinate a funzioni ben più nobili

capitato negli ultimi cinque anni che un'arma classificata dal banco di prova secondo le normative comunitarie non sia stata catalogata dall'istituto nazionale catalogo delle armi nel nostro Paese.

Qui è in gioco l'attinenza di questa norma con il tema del provvedimento, che ha ad oggetto la «proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace».

un argomento che è estremamente delicato e complesso e che sicuramente dovrà essere affrontato, ma che nulla ha a che vedere con l'oggetto del testo su cui stiamo discutendo, cioè la proroga delle missioni Avventurarci oggi in una discussione che riguarda la classificazione o meno delle armi da guerra, il modo in cui queste vengano individuate ed escluse o meno dall'elenco di quelle sottoposte ad un regime giuridico particolare mi sembra obiettivamente una cosa che non ha alcun senso.

visto che il senatore Mazzatorta è certo che ci sarà una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia, aspettiamo che dall'Europa ci venga detto che siamo arretrati rispetto a questo aggiornamento che si vuole proporre oggi, e sicuramente nel giro di poche settimane sarà soddisfatta la volontà della maggioranza. Perché votare?

anche noi rimaniamo particolarmente colpiti dal fatto che, in una legge di conversione di un si introduca un articolo su una materia importante, ma totalmente estranea.

8*‑bis*, che reca modifiche alla legge n. 110 del 1975 sulle armi, senza nessuna organica visione di ciò che si sta facendo. Si interviene in misura pesante su una legge che non c'entra proprio nulla con il decreto. Non si può inserire qualunque cosa in un decreto‑legge

le eventuali correzioni. D'altra parte, non si tratta di una modifica di poco conto: si tratta di un emendamento di circa una pagina e mezza. Si interviene in più punti della legge n. 110 del 1975 in materia di armi. Quindi anch'io ritengo radicalmente inammissibile, signor Presidente, la presentazione di questo emendamento, nel testo corretto proposto dalle Commissioni riunite.

è volto a modificare la discrezionalità assegnata al Ministro della difesa nello scegliere come ridurre i contingenti impegnati nelle missioni all'estero. Pur mantenendo la riduzione di 1.000 unità entro il 30 settembre, questo emendamento prevede che detta riduzione sia da operarsi sul contingente attualmente impegnato in Afghanistan, che dovrà quindi essere completamente ritirato entro il 31 dicembre si svolgesse una riflessione. Intervengo per l'ennesima volta su questo tema, perché l'Italia dei Valori non si stancherà mai di ribadire la propria idea di di gestione della politica estera e di difesa, di partecipazione e di contribuzione al contempo al mantenimento della pace in ogni angolo del mondo. Qui si parla di riduzione del personale, però, dopo tre anni di legislatura, avendo il Governo utilizzato lo strumento del decreto‑legge di solito a cadenza semestrale, e qualche volta anche a cadenza trimestrale o quadrimestrale, credo che la settima o l'ottava volta che ci si trova a discutere di come questa nostra partecipazione alle missioni debba configurarsi. mi riferisco ai continui tagli dei fondi per la cooperazione allo sviluppo, ai quali avete anche, in parte, sopperito, riprevedendo appositi finanziamenti, ma che restano comunque inadeguati e sproporzionati rispetto al costo complessivo sopportato dal nostro Paese per le missioni internazionali.

dell'assegnazione di contributi a singoli programmi specifici (di cooperazione allo sviluppo, ovviamente) in giro per il mondo. Sono note le riserve dell'Italia dei Valori sulla nostra partecipazione militare in Afghanistan. Come sapete, l'Italia dei Valori e per tantissime ragioni: non ultime, le tragedie che ogni giorno, in questo mese, ogni settimana e mezza sopportiamo in silenzio, rispettando il dolore dei familiari. Lo rispettiamo in silenzio, ma con tanta rabbia dentro, che

l'ennesima sfilata di persone davanti ad una bara, che promettono qualcosa che alla fine non mantengono, come non l'hanno mantenuta per 40 volte. colleghi, già personalmente ho sempre avuto difficoltà a capire le spinte federaliste della Lega Nord. Ma che la cooperazione allo sviluppo in Afghanistan debba essere volta al federalismo delle risorse da inviare nelle province afghane mi sembra un po' pericoloso. Le province afghane, al pari, se non più, del Governo corrotto di Karzai, sono rette, come tutti sappiamo, da *leader* tribali, che con una mano prendono i soldi della cooperazione allo sviluppo e con l'altra autorizzano e coprono la produzione di oppio, e vendono, senza neppure troppa furbizia, la vita dei nostri cooperanti, quando non anche dei nostri militari. Signor Presidente, concludo confermando ancora una volta questo nostro dissenso totale a questo

Presidente, noi voteremo a favore di questo emendamento, anche perché, nel dibattito sviluppato in Commissione, abbiamo ricondotto la materia a una scrittura più opportuna. Ricordo, per chi non lo avesse letto, che nel testo originale dell'articolo 9 del decreto varato dal Governo si prevedeva una riduzione dei militari nelle missioni all'estero di 1.000 unità entro il 30 settembre, e di altre 1.070 unità entro il 31 dicembre, attraverso un provvedimento assicurato dal Ministro della difesa. Ebbene, abbiamo sollevato una questione in Commissione. A noi è sembrato che in presenza di una moltitudine

quale missione fosse interessata a tale riduzione ci sembrava una procedura non corretta, soprattutto nel rapporto che si è sempre stabilito tra il Governo e il Parlamento su questa materia.

finalmente introduce in via permanente nel rapporto fra Governo e Parlamento, per le prossime decisioni che riguardano le missioni, l'obbligo del Governo a venire in Parlamento almeno due mesi prima che scada il finanziamento alla missione, per prospettare il suo punto di vista sul quadro generale dell'andamento delle missioni, su quali cambiamenti occorra introdurre e soprattutto quale sia il giudizio del Governo rispetto agli obiettivi che in ciascuna missione devono essere perseguiti.

fra pezzi e parti del Governo il modo in cui dobbiamo stare nelle missioni militari che impegnano il Paese anche nel rapporto con gli alleati, evitando che volta

come è accaduto in questa circostanza e come noi abbiamo provveduto a correggere, e le Commissioni hanno accolto - riducendo prima di 1.000 e poi di 1.070 unità senza che ci sia dietro questa riduzione una discussione sugli obiettivi, sulle finalità e sul ruolo che l'Italia si propone di perseguire con il suo impegno nelle missioni internazionali di pace. *(Applausi dal

li ritiro, anche se voglio fare una difesa linguistica del "nonché", con il quale viene indicata la cooperazione, cioè quell'1,9 per cento attraverso cui il titolo rimane un po' truffaldino ma a fasi inverse.

per il mantenimento in Italia di un polo di eccellenza delle Nazioni Unite, che costituisce un momento importante della presenza e dell'azione internazionale del nostro Paese. La riformulazione proposta dal Governo

avremmo gradito una formula più stringente - a valutare la possibilità di procedere alla ratifica dei principali strumenti internazionali in materia di diritti umani, perché secondo noi solo se si sostituisce alla legge della forza la forza della legge ci sarà in Libia la possibilità di un futuro diverso. Concludo dicendo che è anche molto importante tener presente che ci sono tre mandati di cattura spiccati contro Gheddafi, il figlio ed il capo dei servizi segreti;

Signor Presidente, non intervengo nel merito, perché altri ritengo potranno farlo meglio di me. Vorrei soltanto che si desse conto,

che questo emendamento corrisponde ad identico emendamento, già presentato nella legge sulla semplificazione amministrativa. È la seconda volta, quindi, che si cerca di infilare questa normativa in un provvedimento di legge. Ritengo lo dico

quindi chiedere all'Assemblea di soprassedere alla sua approvazione, perché venga fatta una verifica per capire se si sta trattando di una questione che attiene a licenze, cambio di classifica di armi, oppure ad interessi economici. Credo che questo debba far riflettere il Parlamento: si tratta di materia estranea al provvedimento, che tratta

lascia qualche dubbio; però, devo attenermi alla compatibilità della proposta al testo che stiamo discutendo*. (Commenti dal Gruppo PD).* Devo replicare. Il senatore Zanda ha osservato che questo emendamento è stato presentato in altri provvedimenti: ne prendo atto. A me compete verificare la compatibilità di questo emendamento con l'argomento trattato col decreto.

Non capisco perché non possiamo fare una discussione serena su tale questione e perché siete così nervosi! Dateci la possibilità di discutere: stiamo parlando di un provvedimento importante!

cambiando sostanzialmente la disciplina sull'uso delle armi nel territorio italiano, con la scusa di agevolare il compito della nostra missione all'estero per alcune persone. È una cosa obiettivamente di notevole gravità che, al di là dei profili di inammissibilità, attiene al merito della questione. Non è un atto serio rispetto al provvedimento che stiamo affrontando. Nessuno discute che si tratti di un una materia che, essendo regolata dal testo unico di pubblica sicurezza, che è datato, debba essere adeguata; ma non è questo il modo, né la sede, né la forma attraverso cui possiamo dire quali sono le armi da guerra e quali non lo sono. Lo facciamo inoltre non

vorrei appellarmi a lei, al Governo e alla maggioranza, perché questo non è un provvedimento qualunque;

Per tradizione ormai consolidata, che ha scavalcato anche l'alternanza politica, in questo provvedimento si riconosce la gran parte del Parlamento, al di là degli schieramenti politici. allora che sarebbe una norma di *fair play* parlamentare elementare astenersi dall'introdurre all'interno di questo decreto,

valutazione. Credo che introdurre norme di questo genere metta una parte di questa Aula in imbarazzo, dovendo votare e sapendo di dover votare un provvedimento nel quale riteniamo che la gran parte del Parlamento si debba riconoscere, perché in esso si riconosce la gran parte del popolo italiano.

è destinato alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi ed agli equipaggiamenti dei nostri soldati nelle missioni, per cui la pertinenza, oltre ai profili già illustrati perfettamente e tecnicamente dal relatore Esposito, si lega al fatto del recupero delle risorse. Dove individuiamo queste risorse? Ci sono delle stratificazioni nel nostro ordinamento, delle croste come le abbiamo definite, che non si riesce a rimuovere: una di queste è la commissione di omologazione, che blocca ogni piccola variazione di ogni arma sottoposta al catalogo nazionale, fatto che non esiste in nessun Paese d'Europa.

un prodotto risponde alla legge, ma nel nostro Paese questo *iter* dura mesi, mesi e mesi. Indubbiamente per le imprese - è vero, è anche una questione di interesse economico - ciò costituisce un grandissimo freno. Pensate che un'arma sportiva, soltanto perché muta un mirino, dovrebbe richiedere l'omologazione a questa commissione: è anacronistico, frena l'economia e non si giustifica; inoltre ha grandi costi che è meglio recuperare e destinare alla sicurezza delle missioni dei nostri militari all'estero.

Noi stiamo esaminando un provvedimento che riguarda il rifinanziamento delle missioni delle nostre

che i risparmi conseguenti alle modifiche normative della legge 18 aprile 1975, n. 110, vengano destinati destinati alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi e degli equipaggiamenti impiegati nelle missioni internazionali, non giustifica la pesante modifica apportata

Non vorremmo che un intervento così nobile e così delicato riguardante i nostri militari all'estero venga inquinato da logiche di mercato delle aziende che producono armi. Noi vogliamo separare le due questioni. Non vogliamo che ci si approfitti si approfitti di un decreto firmato dal Capo dello Stato per venire incontro agli interessi di qualche gruppo monopolista! Questo è il problema: non lo votiamo perché non votiamo le porcherie! È evidente che abbia un carattere di opportunità politica la valutazione del Presidente sull'ammissibilità di un emendamento. Mi permetto però di aggiungere anche la nostra voce alla sollecitazione che le viene rivolta. Se è vero, come appare vero, che questo emendamento rientra in un equilibrio politico della maggioranza

che non stiamo ora affrontando, Presidente, un decreto‑legge insignificante per il Paese. Dunque, la riflessione che si impone a mio modo di vedere al Presidente è se questo non comporti che alcune forze parlamentari, che voterebbero a favore del decreto sulle missioni, magari anche superando alcune riserve interne, possano essere indotte - dall'introduzione di materie chiaramente ultronee e che forzano alcune sensibilità - a negare il proprio assenso alle missioni all'estero, poiché il decreto che viene configurandosi non solo assume profili estranei

Si può scegliere di trasformare inopinatamente una materia, che nel tempo e in tutti questi anni si è trattata con grande cura da parte dei Governi che si sono succeduti, affinché avesse il più largo consenso possibile a favore dei nostri militari, a garanzia della convergenza nazionale sulle missioni italiane all'estero, ma si rischierebbe - e ciò va soppesato, signor Presidente, molto seriamente - di danneggiare un bene primario comune per

a constatare che a causa di tale decisione venga meno l'unità nazionale sulle missioni dei nostri militari all'estero, sarebbe davvero una grossa frittata che l'Assemblea del Senato dovrebbe fronteggiare; e penso che sarebbe un pessimo messaggio per il nostro Paese.

Non conosco la norma nelle sue sfaccettature e nelle sue ricadute industriali, e può darsi che sia pienamente legittima e aderente ad interessi del tutto corretti, ma certamente le riflessioni che il collega Tonini, e subito dopo il presidente Rutelli, le hanno molto opportune e dovrebbero ispirare, anche nella maggioranza, quel di più di prudenza e di correttezza nelle relazioni parlamentari per salvaguardare un provvedimento che si inserisce in un clima, che faticosamente si ricerca, di grande rispetto tra le parti quando vi sono interessi nazionali in gioco. Qualche giorno fa abbiamo operato in piena in piena condivisione in una tempistica strettissima per arrivare all'approvazione di una manovra finanziaria difficile e molto delicata. Già c'è questo *vulnus* che riguarda il processo lungo,

intatto il suo valore originario e tutti noi possiamo votarlo serenamente.

tale testo e, gliene devo dare atto, sulla base di una discussione che abbiamo avuto in relazione agli effetti più negativi dell'emendamento aggiuntivo, con particolare riferimento alla modifica dell'articolo 1 relativamente alle armi da guerra. guerra. Non so se questo testo 2 sia stato presentato o debba essere presentato, perché almeno per quella parte, e mi faccio carico di questa situazione (perché se dovesse entrare in vigore in futuro - mi auguro di no una norma di questo tipo creerebbe davvero dei danni nella lotta alla criminalità), se questo testo 2 esiste davvero e viene presentato - e lo chiedo al presidente Bricolo - dovrei dare atto che quanto meno quella parte di pericolosità si cerca di ridurla.

prima presentato anche all'opposizione una possibile riformulazione, che però deve essere integrata con l'emendamento che in questo momento è nel fascicolo.

chiedendo espressamente di posticipare alla fine del calendario, così come da lei comunicato all'inizio di questa seduta (quindi, alla settimana prossima) l'esame del disegno di legge cosiddetto sul processo lungo (a prescindere dalla rubrica che ancora è recata sul frontespizio del provvedimento). Siccome è una richiesta molto seria e poiché riteniamo che i decreti in via di conversione e l'esame e l'approvazione del bilancio del Senato, che è importante in sé ma quest'anno è ancor più importante per tutte le ragioni che conosciamo (tutta l'Italia guarda al suo esame, all'approvazione e agli orientamenti che le due Camere assumeranno su questa materia), sono più urgenti doveroso posporre la discussione di questo provvedimento al quale nessun italiano - o forse due, tre - pensano in questo momento e vogliono che venga esaminato. insistiamo su questo punto, sapendo che il Regolamento prevede tale possibilità.

la conversione anche in termini procedurali che la maggioranza ha voluto offrire all'Assemblea; tuttavia, per le ragioni che sono state abbondantemente espresse sia in ordine al merito che in ordine al metodo,

volto solo a semplificare la vita di tanti piccoli imprenditori che in questo momento lavorano nel nostro Paese, ma andava a supporto anche delle missioni di pace che noi riteniamo importanti. Come Lega Nord abbiamo sottolineato più volte che,

prima di stabilire il programma dei lavori di domani mattina, la Presidenza informa l'Assemblea - come anticipato dal senatore Legnini - che è stata formulata, da parte dei senatori Finocchiaro, D'Alia, Belisario, Rutelli, Pistorio, Zanda, Legnini, Serra e Giambrone, richiesta: «Premesso che il disegno di legge sul cosiddetto processo lungo non presenta carattere di necessità e di urgenza tale da impegnare in via prioritaria l'Assemblea del Senato, si chiede di posticipare la discussione e la votazione del disegno di legge n. 2567 sull'inapplicabilità del giudizio abbreviato per i delitti puniti con l'ergastolo e di porla all'ultimo punto dell'ordine del giorno del calendario dei lavori programmato per le settimane dal 26 al 28 luglio e dal 1° al 4 agosto».

Onorevoli colleghi, comunico che l'informativa del ministro Matteoli sull'incendio alla stazione di Roma Tiburtina avrà luogo giovedì 28 luglio, alle ore 15,30. Seguiranno gli interventi dei Gruppi per cinque minuti ciascuno. **Mozioni, interpellanze